Signora Presidente, la mozione che adesso mi accingo ad illustrare, presentata dal Gruppo del Partito Democratico, ha come oggetto la istituzione di una Commissione speciale con il compito di elaborare testi di riforma costituzionale su tre questioni: la riduzione del numero dei parlamentari, la riformulazione dell'articolo 81 della Costituzione e la questione in relazione alla soppressione delle Province. Spiace che questioni di questa rilevanza non abbiano attirato la presenza in Aula di un più consistente numero di senatori, sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione. Ma tant'è, questa è una delle condizioni di questa fase delle istituzioni!

il potere di stabilirne la composizione sulla base delle designazioni proporzionali dei Gruppi parlamentari. Ed è una facoltà che in passato il Senato ha utilizzato molte volte con competenze, modalità e costituzione molto varie. In taluni casi, le Commissioni speciali sono state costituite per l'esame in sede referente o deliberante di singole proposte di legge, in altri casi di interi *corpus* di atti o di tutte le proposte di legge attinenti a una determinata materia. In altri casi ancora hanno svolto compiti di studio e di approfondimento o anche di semplice espressione di pareri ad altre Commissioni. Anche le modalità con cui le Commissioni speciali sono state costituite sono varie. Alcune volte la costituzione è avvenuta su proposta del Presidente del Senato ovvero - come potrebbe avvenire in questo caso - a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea, di una mozione. Con ciò voglio dire che la prassi parlamentare in questa materia è particolarmente varia sia per le competenze, sia per le modalità di costituzione delle Commissioni speciali. Ma è anche uno strumento che è stato molto utilizzato nella vita del Senato. Con la mozione che stiamo discutendo, i senatori del Partito Democratico propongono la costituzione di una Commissione per l'esame di alcune rilevanti riforme costituzionali, la cui urgenza si è resa evidente nel corso delle settimane quando il Senato ha affrontato l'esame delle misure necessarie per fronteggiare la crisi economico-sociale che sta rischiando di travolgere l'Occidente, l'Europa e, con particolare violenza,

nel mezzo di una crisi di natura soprattutto finanziaria. Ma dobbiamo pur sapere che la sua origine è negli errori e nei comportamenti degli uomini, nelle decisioni sbagliate o addirittura nelle non decisioni delle istituzioni. unanime convincimento che la crisi si possa contrastare e battere solo se, accanto alle misure di contenimento della spesa pubblica e alle misure dirette alla promozione dello sviluppo e della crescita, verranno introdotte modifiche a quegli assetti istituzionali che stanno immobilizzando il nostro Paese. Sappiamo che gli interventi finora disposti dal Governo italiano hanno aggredito in modo molto parziale Tra l'altro è importante ricordare come la recente manovra di ferragosto (che seguiva di poche settimane un altro analogo provvedimento egualmente molto pesante) sia stata emanata dal nostro Governo con un decreto scritto sotto vera e propria dettatura della BCE. Debbo dire che preoccupa che la nostra inazione possa spingere le istituzioni internazionali a proseguire con questa sorta di protettorato e di supplenza non solo del Governo, ma persino del Parlamento italiano. Vorrei che riflettessimo su quanto siano limitate la sovranità e l'autonomia di un Paese, le cui condizioni rendono necessario che le manovre economiche siano dettate da una Banca internazionale, la stabilità politica venga richiesta e sanzionata dalle agenzie di *rating* e che la moralità dei governanti venga richiamata dalla Santa Sede. Sede. Mancano tuttora politiche e programmi per la crescita e mancano le sempre più urgenti riforme del sistema istituzionale, ormai in molti punti palesemente inadeguato. La previsione di una Commissione speciale per l'esame delle più urgenti riforme costituzionali non muta le competenze della la Commissione, al cui lavoro all'iniziativa del presidente Vizzini (che in questo momento, però, discute con il presidente Gasparri, quindi non ha la possibilità di ascoltare quel che gli sto dicendo) gli sto dicendo) si deve la recente e molto positiva accelerazione dell'esame dei disegni di legge riguardanti la riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta di provvedimenti che giacevano dimenticati in Commissione dall'estate 2008 ed oggi, forse anche in vista della possibile costituzione della Commissione speciale, sono stati posti all'ordine del giorno e speditamente esaminati. esaminati. Tutto il Gruppo del Partito Democratico si augura che l'Aula del Senato possa discutere e approvare questa importantissima e attesa misura entro le prossime due settimane. I tempi che viviamo sono tempi speciali nei quali può essere necessario che agli strumenti ordinari vengano affiancati strumenti capaci di maggior efficacia e maggior rapidità di esecuzione. che la Commissione speciale da istituirsi per esaminare le modifiche all'articolo 81 della Costituzione e il nuovo assetto delle autonomie locali connesso all'abolizione delle Province veda la partecipazione dei Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Senato; Senato; una così qualificata composizione potrebbe attribuire particolare efficacia, autorevolezza e speditezza al lavoro della Commissione. Il Partito Democratico crede e difende la natura parlamentare della nostra democrazia e auspica che il Parlamento possa essere la sede nella quale le riforme che servono al nostro Paese vengono proposte, discusse ed elaborate Non sotto la dettatura di altri. Al Partito Democratico non piace che il Parlamento venga ridotto ad organo di mera approvazione di ordini e contrordini voluti ed elaborati altrove, nelle sedi dei partiti, negli uffici legislativi del Governo e persino nelle cene non nella sede istituzionale di palazzo Chigi, ma, come non accade in nessuna altra parte del mondo, in quella privata di palazzo Grazioli. Troppo spesso in questa legislatura il Parlamento ha accettato di svolgere un ruolo gregario, ha rinunciato alle proprie prerogative e alla propria autonomia, ha tollerato mortificazioni e umiliazioni. Penso che il Senato debba saper mostrare al Paese, alla comunità internazionale e ai mercati di voler fare sul serio, di voler riformare senza più alcuna dilazione le istituzioni pubbliche. Penso che dovremmo farla finita con quelle tattiche politiche che pongono obiettivi sempre più vasti e, così facendo, fingono di voler far tutto per poi finire col non far nulla. Perché il Parlamento in tempi di grave crisi possa adempiere alle sue responsabilità di legislatore è necessario che venga messo in grado di utilizzare tutti quegli strumenti che il nostro Regolamento prevede e che sono necessari per risolvere con la maggiore incisività possibile i problemi. In primo luogo, i problemi che attengono all'assetto delle istituzioni. L'antipolitica dilagante, il disprezzo popolare nei confronti di quella che ormai tutti chiamano «casta», la disistima pubblica per le istituzioni, compreso lo stesso Parlamento, sono una conseguenza diretta della delusione dell'opinione pubblica nei confronti delle promesse non mantenute da parte del populismo demagogico con cui l'Italia è stata è stata governata negli ultimi dieci anni. Il discredito del Parlamento deriva anche dalla nostra ormai troppo lunga incapacità a governare i fenomeni e a trovare soluzioni. La proposta di costituire una Commissione speciale, e l'auspicio che ne possano far parte tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato, non è una proposta tattica, né una proposta dilatoria «di opposizione». È una proposta costruttiva che il Gruppo del Partito Democratico avanza all'Assemblea del Senato come contributo a migliorare la qualità del lavoro parlamentare, cioè del nostro lavoro.

del Governo, se non ci trovassimo in un contesto estremamente preoccupante, di crisi economica globale e di crisi politica che è, invece, particolarmente italiana, forse il tema della riduzione del numero dei parlamentari non si sarebbe imposto all'attenzione collettiva come un punto ormai imprescindibile. La riduzione del numero dei parlamentari di per sé è stata anche criticata da molti colleghi sapienti che sono intervenuti nel nostro dibattito in Commissione affari costituzionali perché vi ravvedono un impulso punitivo, un'inefficacia tecnica, una discutibilità nei risultati. Sono stati fatti paragoni con i Parlamenti europei, e molti colleghi si sono esercitati con il pallottoliere

Queste sono discussioni che hanno una loro dignità, ma che oramai in realtà ce l'hanno soltanto in sede accademica: sono discussioni di scuola. Invece noi, la Commissione affari costituzionali e l'Aula del Senato, siamo costretti ad affrontare di petto una congiuntura che forse avvertiamo soltanto quando ci confrontiamo fuori direttamente con i soggetti dell'opinione pubblica, i promotori, i giornalisti, i giornalisti, i cittadini che incontriamo nella nostra vita normale. Qui dentro arriva molto ovattato, attenuato, opacizzato l'impulso del rinnovamento che invece troviamo fuori. È necessario che riflettiamo molto su questa discrepanza di sensazioni. Qui non si avverte l'urgenza, però basta uscire da qua per avere fortissimo il senso di una ragione... Ha ragione, senatore Pardi, però è anche antipatico continuare a interrompere chi interviene. PARDI *(IdV)*. ...di una ragione che non è aritmetica. Qui sembra che noi discutiamo di numeri, ma in realtà discutiamo del destino. La ragione non è aritmetica, è ragione politica. Ci sono cose che il Parlamento non può fare nonostante le aspirazioni demiurgiche; un Parlamento non può stabilire che improvvisamente il processo economico riparte e la società ridiventa fluente, i redditi crescono e le speranze si rinnovano: sono cose che sfuggono. Il Governo e il Parlamento possono aiutare, dare una mano, ma non possono decidere e ottenere un risultato su questo terreno. Il Parlamento, e qui il Senato, può invece prendere di petto il senso della propria responsabilità. Noi siamo oggi obbligati (e se non ce ne rendiamo conto facciamo un errore colossale) a rispondere a una domanda di serietà che ci viene da parte della società, e dobbiamo dare un segno. Può darsi benissimo che la riduzione del numero dei parlamentari possa apparire come un artificio numerico, ma non lo è proprio perché deve riuscire a far capire alla totalità dei cittadini che i sacrifici, i tagli, le rinunce, la sobrietà, che noi chiediamo a tutti, meno che a noi, si rivolgono fin dall'inizio, in un senso quasi ontologico, su noi stessi. Se il Parlamento non trova la forza di far capire fuori che il meccanismo globale della ridiscussione dei principi dell'economia e della politica parte parte da qui incidendo nella carne delle Aule rappresentative, noi risultiamo incredibili. Questo è il punto fondamentale.

una globalità di ragionamenti più ampi; per esempio, hanno ragione tutti i colleghi che dicono che la riduzione del numero dei parlamentari non può essere una cosa a sé stante, che deve essere inserita in un contesto di soppressione delle Province, cui io aggiungerei la riduzione dei Consigli regionali che, come vi è noto, sono dei veri e propri Parlamenti, dispendiosi e gravosi per la comunità intera del Paese. Certamente c'è questo quadro globale, ma noi in Commissione affari costituzionali abbiamo cominciato, giustamente, secondo me, a prendere di petto l'unico argomento che potevamo subito mettere all'ordine del giorno: la riduzione del numero dei parlamentari. dei Valori, ad esempio, propone il dimezzamento, altri propongono diminuzioni meno rilevanti; ma il punto è questo. Se noi ci divincoliamo di fronte a questo dovere e troviamo delle forme per dilazionare questa discussione rischiamo un nostro *default* politico di fronte all'opinione pubblica, di fronte a chi ci ha eletto. Penso che i cittadini saranno capaci di capire il peso della nostra azione soltanto se noi dimostriamo che la nostra azione comincia da noi stessi. Se non facciamo questo perdiamo l'autorità politica che immaginiamo di avere. Per questo motivo, ho ascoltato con sollievo la parte del discorso del collega Zanda in cui ha detto apertamente che la proposta della Commissione speciale non deve confliggere con il cammino intrapreso dalla Commissione affari costituzionali e non rappresenta un espediente dilatorio rispetto a tutta la questione. Questo ci conforta. Noi riteniamo che la discussione in Commissione affari costituzionali su questo tema debba procedere con

il Parlamento, il Senato possono fare per riscattarsi dall'inazione, dalla incapacità di decidere. Non tocco qui gli aspetti generali della incredibilità della politica italiana. Data l'attuale condizione, ormai il Presidente del Consiglio non può più nemmeno andare all'estero, perché non può essere ricevuto da nessuno. La credibilità internazionale di questo Governo è caduta sotto i tacchi. Abbiamo la possibilità di costruire un rinascimento del Parlamento, e questo è un punto di applicazione. Può sembrare modesto, può sembrare numerico: invece, in realtà, è un piccolo passo che ci permette di invertire una tendenza che ormai, negli ultimi tempi, è diventata davvero insostenibile. Perciò il Gruppo dell'Italia dei Valori chiede il voto su una mozione che mette all'ordine del giorno questo tema con la massima nettezza, con la massima semplicità, senza nessun fronzolo, per cominciare un cammino che riconquisti alla Repubblica la dignità della politica.

colleghi, nonostante il bel discorso del senatore Zanda (che ho veramente apprezzato) così come quello del senatore Pardi, l'esito del dibattito odierno mi sembra sia già segnato.

Sono dunque realmente superflue queste mozioni? Se analizziamo la realtà, che è sotto gli occhi di tutti, notiamo che ci troviamo di fronte ad una serie di iniziative scoordinate:

vi è un *referendum* che con ogni probabilità verrà votato nella prossima primavera e che è destinato a cambiare la legge elettorale attuale; vi è un disegno di legge governativo che vorrebbe abolire le Province, ma che in realtà non le abolisce affatto. Ebbene, abbiamo di fronte un anno e mezzo di tempo, ma se non vi sarà un coordinamento tra tutte queste iniziative ed altre ancora, il rischio che salti tutto è sicuramente molto forte. dubbio si avverte la necessità di una proposta coordinata, che reagisca al solito vezzo politico italiano di affrontare le emergenze sotto la pressione dell'opinione pubblica e dei *mass media*, al di fuori di un piano strategico e di una visione sistemica. In realtà, è giunta l'ora di portare a compimento quel percorso di riforme istituzionali la cui esigenza è stata manifestata per alcuni temi già 20 anni fa, innanzi tutto partendo dalla razionalizzazione degli enti territoriali. Ora essa è collegata giustamente alla necessità di ridurre la spesa pubblica, ma tale esigenza non nasce soltanto oggi; sotto la spinta di un'economia dissestata diventa indispensabile, ma essa risponde ad una revisione complessiva dell'ordinamento repubblicano tanto più utile in coerenza con la stessa riforma del Titolo V della Costituzione.

per meglio gestire il progetto federalista senza gravare eccessivamente sul bilancio dello Stato. La fondazione Agnelli immaginava di istituire 12 Regioni, cioè di accorpare le Regioni in 12 macrounità. Peraltro, non dobbiamo dimenticare che in il divieto di istituire Regioni sotto il milione di abitanti, proprio per evitare di frammentare eccessivamente l'istituzione regionale indebolendola

soltanto in attesa dell'introduzione dell'istituto regionale. Le Province dunque erano destinate ad essere soppresse con l'avvento delle Regioni, altrimenti avrebbero rischiato di introdurre una conflittualità tra i due istituti e un doppione non necessario. L'abolizione delle Province determinerebbe a regime un risparmio di circa 3 miliardi di euro. Credo dunque che un'autentica soppressione di tale istituto sia indispensabile sia per fare funzionare meglio il nostro sistema degli enti territoriali sia anche per risparmiare considerevoli risorse. L'accorpamento dei Comuni è stato fatto quasi ovunque: in Gran Bretagna, in Belgio, in Danimarca, in Svizzera; lo si propone per la Francia ed è stato realizzato in Grecia per affrontare il problema del debito greco.

apposito. La riduzione del numero dei parlamentari necessita a maggior ragione di una modifica della legge elettorale, necessaria perché la legge elettorale attuale provvede alla sostanziale nomina di deputati e senatori non dà un adeguato spazio alla voce ed alla libera scelta dei cittadini. D'altro canto, signor Ministro, la riduzione del numero dei parlamentari con questa legge elettorale,

rischiamo di concentrare in pochi soggetti nominati il potere di decidere il futuro di questo Paese. È un meccanismo che si tiene insieme: riduzione del numero dei parlamentari e riforma della legge elettorale devono andare di pari passo.

La revisione del bicameralismo diventa assolutamente indispensabile oggi in un momento, tra l'altro, in cui le decisioni che noi dobbiamo prendere devono essere sempre più rapide e devono essere sempre più puntuali. Non possiamo permetterci più una doppia lettura dei provvedimenti che comporti una perdita di tempo. È chiaro che tutto questo disegno articolato si tiene insieme. necessità di rivedere anche il riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Signor Ministro, credo che questo possa interessarle, perché noi siamo per eliminare il più possibile le competenze concorrenti. che l'introduzione delle competenze concorrenti ha dato luogo a un'esplosione dei ricorsi di fronte alla Corte costituzionale, ad un'incertezza su chi è realmente titolato ad intervenire in determinati settori vitali per lo sviluppo del Paese. anche la revisione dell'articolo 117 della nostra Costituzione dovrebbe essere messa all'ordine del giorno. Riduzione delle spese della politica e revisione dell'articolo 81 vanno di pari passo perché l'obbligo del pareggio di bilancio è indubbiamente un passaggio indispensabile proprio per contenere quelle spese e a sua volta può essere agevolato dalla riduzione dei costi della politica. Infine credo sia arrivato anche il momento di rivedere i rapporti tra politica e magistratura, garantendo una piena indipendenza e responsabilità.

Tutto questo può e deve essere rapidamente affrontato con un organismo ristretto che faccia, entro un mese, entro novembre, da cabina di regia. Riforme così rilevanti, in particolare la riforma della legge elettorale, non possono che essere votate da una maggioranza ampia e non possono essere imposte da una maggioranza espressione solo del Governo. In nessun Paese al mondo la riforma della legge elettorale viene votata con maggioranze ristrette. Sarebbe un precedente importante, invece, se noi riuscissimo ad avviare oggi un dialogo fecondo, un'occasione di confronto che è stata auspicata più volte anche dal presidente Napolitano, ed un dialogo *bipartisan*, costruttivo e aperto, nell'interesse generale del Paese. Proprio per questo noi insistiamo su questa mozione,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel corso dell'estate, esattamente il 25 agosto, da parte del Gruppo del Partito Democratico, in particolare dalla presidente Finocchiaro, fu avanzata pubblicamente la proposta di istituire una Commissione speciale, con l'auspicio che della stessa entrassero a fare parte i Capigruppo del Senato ed altri esponenti che

di accelerare il processo riformatore. In particolare in quella nota si faceva riferimento a tre questioni: l'abbattimento del numero dei parlamentari, la riforma dell'articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio

per non parlare dei provvedimenti riguardanti il federalismo che investono le Regioni e gli altri enti locali.

dicendo letteralmente: «Al di là dello strumento proposto, che non ci sembra il più idoneo» - cito da un'agenzia del 25 agosto - «anche perché in una situazione nella quale l'opposizione è articolata in un numero di Gruppi superiore a quello della maggioranza una Commissione speciale formata dai Capigruppo non sarebbe rappresentativa degli equilibri dell'Assemblea, il proposito di sottrarre all'improvvisazione e alla logica politica di parte materie di rango costituzionale certamente è meritevole di attenzione». inoltre che non avremmo fatto cadere questa sollecitazione politica, al di là dello strumento, che, per le ragioni accennate all'epoca, ci lascia perplessi. Non ci lascia perplessi, invece, la volontà di attuare le riforme; anzi, non solo la condividiamo, ma possiamo dire di avere a nostro merito e a nostro vantaggio numerosi tentativi, taluni anche realizzati. Ricordo, con spirito non polemico ma come semplice registrazione dei che nella legislatura 2001-2006 una maggioranza analoga a quella che attualmente governa il Paese, un Esecutivo guidato dall'attuale presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, portarono a compimento un ambizioso ed importante disegno di riforma costituzionale che investiva molte materie, compresa quella della modifica del bicameralismo perfetto del quale tutti, da decenni, giustamente ci lamentiamo per le sue lentezze e per le sue procedure farraginose, e molte altre materie

di tutto può essere accusata tranne che di inerzia riformatrice. Dopo di che, in base alle procedure che la stessa Costituzione prevede, fu attivato dalle realtà politiche che ieri e oggi

e altre realtà politiche, utilizzando il *referendum* confermativo previsto dalla Costituzione fecero prevalere, in un momento di scarso interesse su quei temi e con una scarsa partecipazione elettorale, il no. Il *referendum* si svolse all'indomani di una prova elettorale che non era stata favorevole al centrodestra, ma questo attiene all'analisi dei motivi per cui quel *referendum* ebbe quell'esito.

in tale direzione. Sappiamo bene che ve ne sono altre, al Senato e alla Camera, presentate da vari Gruppi, e questo ci dà la certezza che quella modifica della Costituzione sarà approvata con un grande concorso di forze e di consensi, come peraltro sta accadendo in altri Paesi europei, in ossequio alle decisioni che l'Unione europea ha assunto e alle quali in termini di politiche

è l'operatività decidente, non dilatoria, su un tema così delicato e urgente che il Governo più volte ha sostenuto di condividere. La maggioranza, ovviamente, è al riguardo, come su tutto il resto, in sintonia con il Governo, però ha anche una sua autonoma rappresentazione e presenza nel dibattito, a maggior ragione laddove si interviene sulle riforme costituzionali e del Parlamento,

che il Governo ha presentato - in questo caso posso dire la maggioranza, perché c'è stato anche un confronto politico, come è evidente che sia - un disegno di legge costituzionale di riforma più complessiva. Il Governo ne ha discusso

e attiene anche al numero dei componenti delle Assemblee. Non voglio inoltrarmi in altre discussioni complesse. Ieri, in sede di Conferenza dei Capigruppo, abbiamo parlato di questi fatti, ma è l'Aula il luogo di decisione e le Commissioni il luogo dove formare la volontà. ieri - mi pare il senatore Rutelli - ha ricordato che adesso ci sono anche i *referendum* - non ho capito se li ha citati in modo positivo o negativo - sulla legge elettorale

arricchite dalle proposte e dalle discussioni svolte nel frattempo. Di fatto, non riproponiamo i testi del 2006. Mi auguro che il disegno di legge complessivo del Governo possa essere rapidamente discusso al Senato, arricchito e modificato così come il Parlamento, a cominciare dal nostro Gruppo, riterrà di fare per la riduzione dei parlamentari proceda con rapidità nella Commissione affari costituzionali, così come il presidente Vizzini e altri colleghi con caparbietà lo stanno portando avanti.

con una eterogenesi dei fini (perché non era questo lo scopo della proposta), rallenterebbe il processo riformatore avviato. Invece di accelerare, come sembrerebbe all'esterno, dove l'istituzione della Commissione di decidere, in realtà rallenteremmo, ma non tutti all'esterno hanno il dovere di comprendere le nostre procedure parlamentari, a volte complesse. Non rallentiamo l'*iter* in atto, sospendiamo la votazione su questo strumento per non bocciarlo e tenerlo come uno strumento di riserva: qualora noi stessi si dovesse certificare davanti alla pubblica opinione - non è che il Parlamento svolga in clandestinità le sue attività un rallentamento, una stasi, una inerzia nell'attività riformatrice, avremmo uno strumento di riserva da utilizzare. Non bocciandolo oggi lo preserviamo come una sorta di estintore dietro il vetro, per cui si rompe il vetro e si prende lo strumento che può aiutarci a risolvere il problema e a realizzare le riforme. Questo è il senso della nostra proposta: evitare che si rallenti l'*iter* delle riforme. Siamo impegnati, come Gruppo parlamentare, in particolare al Senato, su tutte le questioni che ho richiamato e che anche furono richiamate nel corso dell'estate, a lavorare alacremente e celermente, e ben vengano

La prima precisazione riguarda la natura dello strumento Commissione speciale. Il senatore Gasparri l'ha paragonata ad un estintore che sta dietro il vetro: ebbene questo non era il tipo di strumento che abbiamo proposto. Noi abbiamo

il senatore Gasparri quando ricorda che il Governo ha presentato pochi giorni fa una iniziativa sulle autonomie e sulle province: ricordo però che il Partito Democratico un disegno di legge costituzionale su questa materia l'ha presentato da anni. Ha ragione il presidente Gasparri - e l'ho fatto anch'io - a dar atto alla 1a Commissione di avere rapidamente istruito, negli ultimi trenta giorni, i disegni di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari. Ricordo, però, e l'ho già ricordato che i disegni di legge su questa materia giacevano in Parlamento da anni sono stati portati all'esame della Commissione e istruiti con questa velocità quando è stata annunciata la presentazione della proposta della Commissione speciale.

noi dobbiamo impegnarci affinché i provvedimenti che presentiamo e che sono necessari al Paese vengano esaminati e approvati in tempi ragionevoli. È questo il motivo per il quale ho chiesto (e mi aspetterei una risposta, e mi rivolgo anche al presidente Vizzini) Vizzini) che il disegno di legge, sul quale all'unanimità la 1a Commissione ha concordato, sulla riduzione del numero dei parlamentari venga in Aula nelle prossime due settimane.

che si chiamava, anche nel 2008, Silvio Berlusconi. Berlusconi, in modo esplicito e diretto, lo ricordate tutti, ha annunciato che questo Governo si sarebbe mosso con una grande attenzione nei confronti dell'opposizione e che per le riforme sarebbe stata ricercata la massima coesione nazionale possibile. Finora, però, di questo spirito, sul quale voi avete concesso la fiducia a Berlusconi, non si è visto nulla! Quindi, adesso annunciate riforme! Adesso il Governo, e il ministro Calderoli, presentano riforme. Ma come volete farle le riforme? Con uno spirito di condivisione, oppure pensate di poter cambiare la Costituzione della Repubblica da soli?

il senatore Valditara, le riforme elettorali, le riforme delle istituzioni e, a maggior ragione, le riforme della Costituzione si fanno insieme.

Signora Presidente, se l'intento dei presentatori di questa mozione era quello di accelerare l'*iter* del disegno di legge sulle riforme istituzionali, possiamo dire che questo obiettivo, di fatto, è stato è stato raggiunto e, dunque, anche noi concordiamo con quanto annunciato dal presidente Gasparri, cioè sull'accantonamento momentaneo del voto su questa mozione. Ringraziamo comunque i colleghi del Partito Democratico per il contributo che hanno voluto dare su questo argomento. Ricordo però al senatore Zanda che noi queste riforme istituzionali le vogliamo fare, e lo abbiamo sempre detto. E quando ci siamo mossi sulle riforme in Parlamento, lo abbiamo sempre fatto con le opposizioni, aprendo un grande dialogo con le opposizioni. Ricordo al senatore Zanda che gli unici che hanno cambiato la Costituzione in questo Paese

è partito l'*iter* di questa grande riforma. Il Governo ha già votato e varato, dunque, una riforma complessiva delle istituzioni di questo Paese

più moderna in grado di dare risposte ai cittadini) a parole sono tutti favorevoli, vedremo il contributo che daranno i Gruppi, non solo nello scrivere il testo, nell'approfondirlo e nel migliorarlo, ma anche nel dare quella velocità necessaria per arrivare il prima possibile a questo tipo di riforma. al merito della istituzione di questa Commissione: si rischiava una sovrapposizione - è inutile negarlo, senatore Zanda

negli spazi liberi lasciati dalle Commissioni permanenti: i commissari delle Commissioni permanenti sono, infatti, i medesimi delle Commissioni speciali. Dunque, di fatto lavorano molto spesso male. Non solo: sarebbe stato anche un costo aggiuntivo. Bisognava eleggere un nuovo Presidente, due nuovi Vicepresidenti, due nuovi Segretari. visto che questo tipo di Commissioni in passato hanno sempre fallito il loro obiettivo; anzi, hanno contribuito ad allungare i tempi di discussione invece che ridurli. Dunque, è giusto per ora accantonare questa proposta, che comunque viene congelata e tenuta solo come *extrema* *ratio*, mentre è giusto invece affrontare direttamente, nella Commissione di merito, questo provvedimento guardandoci tutti negli occhi

queste riforme, fondamentali per il Paese, e starà alla nostra responsabilità se riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Signora Presidente, colleghi, la crisi economica del Paese e della politica, che ci riguarda tutti, e di cui abbiamo parlato anche in coda ad una delle recenti recenti discussioni in quest'Aula, richiedono effettivamente risposte veloci. Le richiedono sui vari settori anzidetti: sul settore economico per rilanciare l'economia, ma anche sul settore delle istituzioni, che sono purtroppo pesanti e lente e non rispondono più ad esigenze moderne. Per tutto questo, i progetti sono molto ampi ed il Governo

È vero - ne do atto anche al presidente Gasparri - che ci sono vari progetti. Ed è vero che anche da parte dell'opposizione sono sostenuti: ma poi i nodi vengono sempre al pettine! Abbiamo incardinato varie riforme, che poi si fermano perché manca la decisione politica di maggioranza su come nel dettaglio articolare le varie proposte. È questo il punto: facciamo l'esempio della riforma costituzionale.

Avevo anche l'onore di avere proposto per primo il testo di riforma costituzionale, che è diventato il testo base in Commissione, è stato praticamente portato a compimento, ma il

il ministro Calderoli, e cioè che prima della legge elettorale si devono fare le riforme. Mi va anche bene, però allora si devono affrontare le riforme, non si deve stare fermi.

varie modalità e soluzioni, che spaziano da 380 membri complessivi, tra Camera e Senato, a 758 membri, con una riduzione un po' più debole.

iniziativa ha provocato un'immediata risposta da parte del presidente Gasparri, che ha sottolineato che la volontà politica c'è. Di questo prendiamo atto. Naturalmente, sono anch'io per la sospensione dell'esame

a una non soluzione, poiché l'unica Commissione speciale che può essere insediata per affrontare questo tema è una Bicamerale di rango costituzionale,

Una parola sulla riforma bocciata dal *referendum* del 2006, che viene qui molto lodata.

anche rappresentativi delle Regioni e pertanto dando più spazio anche alla rappresentanza della popolazione *in loco*. Però devo dire già detto qui in Aula facendo arrabbiare a suo tempo l'onorevole Bossi - che questo purtroppo è stato uno sforzo bloccato, uno sforzo con ottimi intenti da parte della Lega che si è contrapposto però, nello stesso Governo di centrodestra, alle tendenze di allora di Alleanza Nazionale e della Casa delle Libertà, che l'hanno frenato. Cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori un Senato composto da membri che avevano diritto di voto e da altri membri, delegati dalle Regioni, che non avevano diritto di voto;

non solo questa. Questa va fatta con urgenza e con precedenza, perché se si carica troppo il mulo naturalmente quello non riesce in tempi brevi a risolvere il problema.

che non dà spazio agli elettori; è una delle grandi cause della crisi della politica e delle accuse che vengono mosse a noi parlamentari. Infatti, come si sa, in pratica il Parlamento è eletto da pochi vertici pochi vertici dei partiti, eccezion fatta (lo devo dire non per lodare la nostra terra, ma perché abbiamo mantenuto il Mattarellum,, almeno per il Senato) per la Regione Trentino-Alto Adige.

questa immagine, che noi abbiamo interesse di risollevare nuovamente, non per noi personalmente, ma per la difesa delle istituzioni e di questo Parlamento, che deve rimanere il luogo della rappresentanza del popolo. Pertanto, signora Presidente, ringrazio per lo sforzo dei colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, che hanno messo in evidenza l'urgenza di questi temi; concordo, però, con la soluzione proposta di accantonare

Presidente, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti portando le loro argomentazioni, da ultimo il collega Peterlini che coerentemente esprime la sua passione, il suo convincimento. Anche alla presenza del ministro Calderoli, vorrei che ci capissimo, Presidente, su cosa comporta la nostra decisione. Noi abbiamo considerato con favore l'iniziativa della presidente Finocchiaro e del Partito Democratico di definire una sede ristretta nella quale verificare ciò che il collega Zanda ha ripetuto poco fa, ovvero se ci sono le condizioni perché nella parte finale della legislatura si addivenga a delle riforme condivise, essendo chiaro - credo - a tutti i colleghi che è impossibile immaginare un percorso di riforma nell'accidentata condizione della politica a maggioranza, come in parte sembrava accennare - e questa non è una *new entry* - il collega Gasparri, e come in generale, nello schieramento di posizioni di partito e di Gruppo, sembra affacciarsi quotidianamente nel dibattito politico. L'argomento che vorrei sottoporre alla Presidente e ai colleghi è il seguente. sospensiva proposta dal collega Gasparri comporta un rinvio *sine die*, questo contraddice completamente il senso del dibattito svoltosi fin qui, incluse le posizioni espresse dal collega Gasparri.

però fu una coalizione di cui ho fatta parte a varare la modifica del Titolo V. Ebbene, dieci anni dopo dobbiamo essere in grado di valutarne inadeguatezze e falle

Quarto tema: il deferimento a organismi terzi delle decisioni di autorizzazione a procedere (è un tema maturo, lo abbiamo visto, e riguarda sia il Parlamento sia il Consiglio superiore della magistratura). Infine, la modifica dell'articolo 81 della Costituzione. del Presidente del Gruppo del PdL: cercare di uscire dall'ipocrisia. Faccio un esempio con riferimento alla proposta che il collega Belisario Collega Belisario, se lei propone di assegnare, al di fuori di un percorso condiviso,

dicendo che siamo alla più perfetta realizzazione della massima di La Rochefoucauld che diceva che l'ipocrisia è un omaggio che il vizio - e qui non mi riferisco al collega Belisario - rende alla virtù.

Se, per caso, venisse accolta, senatore Belisario, la sua proposta di varare subito la riduzione del numero dei parlamentari,

Quindi, a legislazione elettorale vigente, lasceremmo la previsione della nomina e non dell'elezione dei parlamentari, modificando la Costituzione quanto al loro numero.

dichiarare costituzionalmente ammissibile la richiesta di *referendum*, alla luce della propria giurisprudenza - si troverebbe nell'assoluta impossibilità di dichiarare legittimi i *referendum* poiché il Parlamento avrebbe già deciso di modificare la composizione del Parlamento stesso, riducendolo a 400 e a 250 i parlamentari. Siamo al paradosso dei paradossi, perché chi propone i *referendum* per modificare la legge elettorale e riprodurre il Mattarellum vuole mettere contemporaneamente in atto un meccanismo che vanifica lo stesso *referendum* che ha promosso. In questo

non si può fare finta di mandare avanti in parallelo quattro o cinque provvedimenti di modifica costituzionale, tutti destinati ad infrangersi

Altrimenti, ci si ritrova in Aula entro la fine di ottobre per approvare l'una o l'altra mozione o comunque un testo importante e significativo per tutta l'Assemblea del Senato.

non si convinceva di come poter essere contento, visto che la sua prima proposta riguardava l'istituzione di una Commissione speciale che discutesse della riduzione del numero dei parlamentari, era probabile che questa fosse un'autolimitazione prodromica alla sua proposta. a quest'ora della mattina il numero dei parlamentari sia aumentato indica che il dissenso alla sua stessa proposta inizia ad aumentare. In questo senso, il dissenso

vorrebbe che l'articolo 1 della nostra Costituzione fosse modificato e dicesse - argomento richiamato dal senatore Rutelli - che la nostra

se, contemporaneamente, non si parla della modifica e della riforma della forma di Stato e della forma di Governo? Che significato ha parlare di un Senato fatto da cento senatori con una Commissione bilancio che, a quel punto, sarebbe composta da dieci senatori, e quindi con un bilancio federale approvato da sei senatori su dieci? Se quello così configurato è un Senato che si contrappone tramite *checks and balances* a una

si modificò la legge elettorale e si fece il Mattarellum, nell'impossibilità allora di modificare la forma di Governo, si introdusse una legge elettorale che proiettava l'Italia verso il bicameralismo e verso il presidenzialismo (cercate di ricordare che l'intenzione di Segni doveva essere quella di eleggere il sindaco d'Italia). E così Fini, Casini e tutti noi cercammo di portare avanti questa possibilità di modifica, ma poi non se ne fece nulla. Oggi, il sistema proporzionale, la legge del 2005, non va bene perché noi non siamo né una Repubblica presidenziale né una

significato. Io ad esempio continuo a dire - ne ho già parlato, e il senatore Zanda lo ricorderà, e lo ha detto il senatore Viespoli già a luglio - che la fine di quest'anno e la fine della legislatura avrebbe dovuto essere una stagione di riforme. Ne ho già parlato dicendo che secondo me, oggi, una Commissione parlamentare ha il suo grande significato, in specie se venisse presieduta da un autorevole esponente dell'opposizione, così come lo fu la Bicamerale del 1997-1998. Quest'ultima fallì non già per per Berlusconi, ma perché la divisione all'interno dell'opposizione non consentì di arrivare al punto sperato, e cioè ad una Repubblica che avesse un'autorevolezza e una rappresentatività all'esterno e che, nonostante il

che sappiano di cosa si parla. Ad esempio, lei, senatore Calderoli, perché vuole fare la modifica della forma di Stato e della forma di Governo seduto sui banchi del Governo? Perché non presiede questa Commissione? Perché non rinunciamo a un'opera che viene calata dell'alto, dal Governo. nelle Commissioni? Perché non ne parliamo e non lo

Lo dico perché, rispetto a tutti i temi di cui si è parlato, il problema principale che resta, nonostante le dichiarate volontà di tutti di affrontare

approvata in Commissione alla Camera e poi rinviata in Commissione: temo che avrebbe avuto un esito ben diverso se fosse stata esaminata dal Senato.

mentre al Senato è in corso la discussione sui disegni di legge relativi alla riduzione del numero dei parlamentari, così come è già stata avviata la discussione, che secondo me dovrà essere riaffrontata, sulla riforma elettorale. Il 22 luglio il Governo ha approvato la riforma complessiva della Costituzione, che non tocca alcuno di questi temi e il 14 settembre ne ha dichiarato l'urgenza. Proprio nella giornata di lunedì ho riferito al Presidente della Repubblica i contenuti di quella riforma, anche rispetto agli aggiornamenti che si erano svolti nel corso del tempo. Al di là delle sue prerogative e dei tempi

esclusivamente per un determinato disegno di legge. Quindi, la volontà di caratterizzare politicamente e dar maggior peso alla Commissione nell'esame della Costituzione con la presenza dei Capigruppo può essere ottemperata utilizzando il Regolamento

ci si dà due mesi di tempo a conclusione dei quali si verifica se si è concluso l'esame in Commissione e si è in condizione di andare in Aula. Diversamente, qualunque altra strada può essere affrontata e discussa,

Senato - come risulta in quest'Aula, ma credo lo sia anche alla Camera - perché non dedicare due mezze giornate alla settimana, ad esempio il martedì mattina ed il giovedì,

cui credo che, se questa sarà la volontà, potremmo approvare la riforma costituzionale e, se lo deciderà il Parlamento, dopo i primi

la natura dello Stato e del Governo e la Camera e il Senato saranno due cose diverse, nel senso che saranno due Camere specializzate in cui ciascuno svolga il proprio lavoro e non le stesse cose, necessariamente anche il meccanismo elettorale avrà una natura diversa.

unanimità. Quindi, mi avvicino a questa discussione con questa disponibilità, la disponibilità di chi però le riforme le vuole fare veramente: da una parte e dall'altra.

vanno nella stessa direzione. È emersa anche la perplessità che un rinvio di questa materia possa nascondere

materie comprese dalla senatrice Finocchiaro nelle competenze della Commissione sia effettivamente andato avanti, e quindi ribadire la giustezza della sospensione. Potremo però pubblicamente riconoscere che il nostro intendimento in buona fede non ha avuto un seguito e la Commissione diventa a quel punto un motivo differente di necessità e di sprone per il Parlamento e il Governo. questo per raccogliere le indicazioni emerse dal dibattito e per testimoniare che non esiste alcuna volontà di sospendere per prendere tempo o per non affrontare questioni

Presidente, ho chiesto di intervenire innanzitutto per ringraziare il ministro Calderoli per l'impostazione e il taglio della sua riflessione e anche per aver sottolineato

A me pare che quanto affermato dal ministro Calderoli non sia in contraddizione con la proposta del senatore Quagliariello di chiusura di questo dibattito.

organicità alla riflessione sulle riforme. L'estrapolazione del tema della riduzione del numero dei parlamentari è sbagliata dal punto di vista sistemico, oltre che da quello delle scelte politiche e di cambiamento, perché è giusto partire dalla riforma e dal riassetto costituzionale, dal superamento del bicameralismo e, consequenzialmente, addivenire all'assetto dei due rami del Parlamento e alla definizione della legge elettorale. Credo che questo si possa fare,

mi pare vada in una direzione che è condivisa, cioè: non c'è il ritiro di una mozione, c'è una mozione che vuole essere un indicatore di verifica del lavoro che viene svolto su questi temi.

in ordine al disegno di legge costituzionale: «Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori» Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

nella discussione che si è svolta fino adesso perché la richiesta da me formulata nella seduta di ieri trae proprio origine dalle lungaggini, forse anche da una chiara assenza di volontà politica di realizzare le riforme.

che sentiamo parlare di riforme epocali: di cambiamento della forma di Stato, di una revisione del bicameralismo, della soppressione di enti inutili. Ovviamente nulla: soltanto parole, probabilmente chiacchiere.

si parla di legge elettorale solo perché abbiamo raccolto le firme per stimolare un ragionamento, ma considerando quello che è successo finora riteniamo che

e ci sono volute ben oltre 500.000 firme per rimettere in moto la discussione. L'abolizione delle Province altro inganno per gli italiani, ma anche su questo tema nei prossimi giorni riverseremo centinaia di migliaia di firme, per dimostrare come la

Invece, la proposta Calderoli le cancella per un verso e poi le trasforma in strani enti, in strani mostri regionali. Chi

non il centrosinistra, ma il Paese e gli italiani hanno bocciato, perché era un pessima riforma della nostra Costituzione. Era un grimaldello che faceva saltare tanto di quello che i nostri Padri costituenti avevano formulato. Ecco perché per vedere fino a che punto le chiacchiere continuano a girare in quest'Aula. ringrazio il presidente Vizzini e la 1a Commissione per il lavoro che sulla riduzione del numero dei parlamentari stanno facendo. Ma ciò non basta:

piccoli passi, anche partendo dalla riduzione del numero dei parlamentari, noi diciamo agli italiani tante grosse sciocchezze.

e illustrata dal collega senatore Pardi. Vogliamo cercare di partire veramente. Portiamo il provvedimento in Aula e cominciamo a confrontarci con chi davvero vuole la riduzione del numero dei parlamentari, senza nasconderci

rincorrere gli *input* che possono venire dalla folla, dalla gente, da coloro che ormai vivono quasi esclusivamente dell'antipolitica e dell'antiparlamentarismo.

riteniamo di dover seguire, con la serietà che tutti quanti noi abbiamo nell'impegno parlamentare, l'*iter* corretto che a noi pare stia seguendo la 1a Commissione affari costituzionali, non solo il Presidente, ma credo tutti quanti i colleghi di tutti i Gruppi si stiano spendendo in maniera veramente seria ed adeguata su un tema

perché delle due l'una: vogliamo dare una risposta alla folla che assedia il Parlamento? Allora oggi le diciamo che vogliamo ridurre i parlamentari e seguire una procedura d'urgenza che che non riveste i caratteri dell'urgenza, dal momento che già se ne sta abbondantemente parlando in Commissione affari costituzionali. Altrimenti possiamo dire alla gente, con maggiore responsabilità, che vogliamo fare una riforma,

razionalità un disegno di legge costituzionale rispetto al quale individuiamo una serie di risparmi, non sui costi della politica e neanche sui costi della democrazia. Qui dobbiamo cominciare ad intenderci su quanto costa la cosiddetta politica e quanto costa la cosiddetta democrazia e, per dirla una volta per tutte, quanto ci è costata quella forma di istituzionalizzazione dell'assemblearismo dell'assemblearismo venuta dopo il Sessantotto, quando tutti dovevano partecipare, e partecipare con alcune forme istituzionalizzate e regolarmente ben retribuite da parte dello Stato. Quindi oggi ci troviamo di fronte ad un pullulare di soggetti che costano e che

Si andrà a votare in Molise tra qualche giorno. Il Molise conta 360.000 abitanti, meno della mia Provincia di Lecce. Oggi non dico che voglio abolire la Regione Molise, ma che semplicemente si può discutere sul

delle unioni dei Comuni, perché gli 8.000 Comuni, di cui tantissimi inferiori addirittura ai 1.000 abitanti, rappresentano un costo non più sopportabile in una democrazia che deve rispondere ad esigenze di partecipazione, ma anche in uno Stato che deve

senatori, riforma che partorirebbe veramente ben poca cosa; piuttosto, che senso ha oggi, in un'Italia federale, avere un certo tipo di Senato? Noi, per esempio, ipotizziamo un Senato delle autonomie, con rappresentanze che vengano dalle Regioni e dagli enti locali, escluse naturalmente le Province, visto che a queste oggi non riconosciamo una funzione essenziale (che peraltro non hanno, non avendo neanche avuto le deleghe dalle Regioni, e quindi non non assolvendo neanche i compiti che attualmente dovrebbero regolarmente svolgere). In tutto questo naturalmente si inquadra anche la riduzione del numero dei parlamentari. senso ha allora, collega Belisario, invocare oggi l'urgenza su un tema che già è in discussione e giocare di rimessa rispetto invece ad un progetto che ha veramente una grande ambizione, quella di poter modernizzare finalmente lo Stato e di essere anche coerenti nel momento in cui facciamo una produzione legislativa che non può essere così frammentaria e frammentata, semplicemente perché dobbiamo rispondere alla folla che sta assediando Montecitorio?

Signor Presidente, credo che l'errore più grossolano che il Parlamento possa fare è quello di

talvolta speculatori, che parlano di casta, che infieriscono sui parlamentari.

stiano facendo un lavoro sacrosanto e utile. Naturalmente, se parliamo di riforme costituzionali l'attenzione deve essere ancora

errore grossolano. Stiamo parlando di riforme di Stato e di Governo, di riforme costituzionali: valutiamole, la fretta è assolutamente controproducente rispetto ad ogni cosa positiva. il collega Ferrara: ma di che parliamo se non vediamo le cose a largo raggio, se non vediamo prima una riforma dello Stato, come lo vogliamo impostare, come vogliamo modificare le Regioni, come vogliamo ridurre i Comuni, come vogliamo

periodo unificando una serie di disegni di legge, che hanno portato ad un intendimento comune secondo cui va ridotto il numero dei parlamentari, vanno abolite le Province va ridotto il numero dei consiglieri regionali. Un buon lavoro. questo intervento che dissocia il disegno di legge dell'Italia dei Valori dagli altri, questa richiesta di

in Aula molto presto. Quindi, francamente mi sforzo di capire la richiesta dell'urgenza e l'estrapolazione dal contesto di un solo disegno di legge; ma tant'è. Ho l'impressione che si voglia mettere il cappello sul provvedimento di riduzione del numero dei parlamentari e si voglia dire: siamo stati noi ad aver ottenuto questo

È un atteggiamento strano. Io non posso sottovalutare il fatto che si voglia dare urgenza a tale questione, anche se ritengo che comunque ci sarebbe stata questa urgenza. Mi auguro però che questa urgenza, se dovesse essere approvata la richiesta dell'Italia dei Valori, non porti a confusione; una confusione che - come ho detto prima - scaturisce dall'urgenza.

Signor Presidente, colleghi senatori, del giorno. Mi viene da citare una frase celebre ai componenti del Gruppo Italia dei Valori: se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica (federale, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Ho il sospetto, infatti, caro senatore Belisario, che il celeberrimo monito rivolto dall'intraprendente Tancredi al principe di Salina calzi perfettamente alla richiesta con la quale si avanza un estemporaneo, obsoleto - dico io - e, a conti fatti,

appare condivisibile in linea di principio, ma a ben vedere è più opportunistica che opportuna, poiché è controproducente agli effetti della stessa finalità finalità dichiarata. Vorrebbe dire ricominciare da capo con la discussione generale, con la presentazione degli emendamenti e così via. Voglio aggiungere che questo è un dispetto

controreplica alla proposta della mozione a firma Finocchiaro ed altri, che abbiamo discusso ampiamente in precedenza. Insomma, la 1a Commissione all'uopo è già impegnata. senatore Serra ha ricordato che il 30 settembre scade la data per la presentazione degli emendamenti, dopo di che si potranno tirare le prime conclusioni. È stato avviato l'esame di proposte di legge per la riduzione del numero dei parlamentari; fra queste n'è anche una della Lega Nord, che ha proposto 250 senatori e 250 deputati. Pensiamo ad un Parlamento con 500 membri, come ha sottolineato il Ministro per la semplificazione, il quale si è detto convinto di procedere e di avere la possibilità di mandare in porto le riforme costituzionali, e dunque varare la nuova forma di Stato e la nuova forma di Governo entro il 2013.

questa circostanza dovrebbe indurci ad operare tenendo conto della necessaria celerità, ma mi sembra che qui tutti stamattina lo abbiamo ampiamente confermato. Ritengo che la chiarezza delle attribuzioni sia la via maestra; d'altronde abbiamo avuto dei precedenti e dei trascorsi non precisamente incoraggianti che ci inducono a invocare con decisione e senza tergiversare la strada della linearità e a nutrire un ragionevole scetticismo dinnanzi alle proposte di chi oggi si dimostra più realista del re riguardo al ridimensionamento della rappresentanza parlamentare. In conclusione, signor Presidente, non ci sentiamo di condividere la proposta formulata

di riduzione dei costi inutili della politica, rivendicazioni sollecitate dai cittadini ben prima che la contingenza economica internazionale le rendesse non più eludibili.

eviterei di fare una lettura quasi sovversiva del nostro Regolamento. Abbiamo invocato il richiamo ad un istituto previsto dal nostro Regolamento quando si ritiene che un voto dell'Aula possa svolgere una funzione sollecitatoria rispetto a dei provvedimenti che si ritengono importanti per il Paese. Peraltro, il Regolamento stesso stabilisce in cosa si traduce la declaratoria di urgenza votata dall'Assemblea,

il primo della classe

riteniamo noi che 630 deputati siano forse eccessivi per il nostro Paese, così come 315 senatori? Sul fatto che è un numero

Noi sappiamo che i termini sono sempre molto elastici da noi, nel senso che sono sempre ordinatori e mai

sia un atto sovversivo. Per favore, dite se volete farlo oppure no; se volete chiacchierare e non farlo - perché, alla fine, probabilmente questo è il vostro obiettivo - affermatelo chiaramente.

forse altri avranno bisogno di alcuni mesi di riflessione, ma è un problema loro. Noi abbiamo normali capacità intellettive e riteniamo che in alcuni giorni questi problemi possano essere

Pochi giorni dopo l'inizio della legislatura, i senatori del Partito Democratico (primo firmatario il nostro vice presidente, il collega Zanda) hanno depositato un disegno di legge costituzionale che prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari,

Poche settimane dopo, il collega Benedetti Valentini, iscritto al Gruppo del PdL,

e subito dopo ripresentato; anche il disegno di legge della Lega Nord prevede una sostanziosa riduzione del numero dei parlamentari. Un analogo provvedimento è stato presentato anche dai colleghi dell'UDC da ultimo, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato un apposito disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari; per essere obiettivi, ricordo che i senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori avevano previsto una riduzione del numero dei parlamentari in un più organico

l'inizio della discussione sull'argomento. Analoga cosa abbiamo fatto in Commissione affari costituzionali chiedendo al presidente Vizzini e all'Ufficio di Presidenza di calendarizzare la discussione di legge. In Commissione affari costituzionali, nel mese di luglio - questo particolare il collega Zanda non l'ha ricordato nel suo intervento, ma ci tengo a precisarlo

a un esame dei disegni di legge che riguardano esclusivamente la materia della riduzione del numero dei parlamentari, stralciando l'esame da quello delle più complessive ed importanti questioni che riguardano riguardano altri aspetti della riforma costituzionale: ad esempio il superamento del bicameralismo, la questione relativa alla legge elettorale (pur non materia strettamente costituzionale). C'è stato un dibattito acceso in Commissione - il collega Benedetti Valentini lo ricorderà, poiché in quel momento presiedeva la Commissione - nel corso del quale si sono scontrate originariamente due posizioni: quella dei colleghi di maggioranza, che prevalentemente ritenevano opportuno discutere di tale argomento nel quadro più generale della riforma costituzionale o che fosse preferibile aspettare un intervento del Governo in materia, e quella dei colleghi del Partito Democratico,

(o perché si tratta di leggi costituzionali o perché si tratta di materia attinente all'attuazione delle norme costituzionali), ha proceduto a nominare due colleghi relatori: un senatore che fa parte di un Gruppo di maggioranza e un senatore che fa parte di un Gruppo dell'opposizione.

Il presidente Vizzini ha dato incarico ai due relatori di predisporre un testo unificato: con uno spirito di collaborazione che non è frequente

Abbiamo trovato un'intesa che si è collocata in una posizione intermedia, per quanto riguarda il numero dei parlamentari, tra la posizione espressa dal Partito dal Partito Democratico e dagli altri Gruppi e quella esposta nel disegno di legge del collega Benedetti Valentini: l'ipotesi su cui abbiamo lavorato prevede la riduzione del numero dei deputati a 450, e la riduzione dei senatori a 250.

e con l'intervento importante del Presidente Vizzini, saremo in grado in poche sedute, se ci saranno le condizioni, di chiudere l'esame del disegno di legge e di licenziarlo per l'Aula in modo tale che -

Democratico voteranno, evidentemente, ed egualmente, a favore, avendo però precisato bene quali sono i termini della questione. Ritengo che se la volontà politica prevarrà, come è accaduto in questi primi giorni di settembre, di settembre, sicuramente in Commissione licenzieremo rapidamente il testo e l'Aula lo potrà esaminare quanto prima. *(Applausi Signor Presidente, colleghi senatori, abbiamo appena concluso una discussione sull'ipotesi di istituzione di una Commissione che nasce dalla volontà

tende invece ad isolare il tema della riduzione del numero dei parlamentari. È un'iniziativa legittima, fatta alla luce del Regolamento, quindi vorrei rassicurarla, collega Li Gotti, sul fatto che non esiste nessuna volontà e nemmeno nessuna intenzione di criminalizzarla né di smontare il Regolamento.

del numero dei parlamentari inerisce innanzitutto il problema della rappresentanza che, come lei sa e mi insegna, è il fulcro stesso del parlamentarismo. Non è un tema che può essere ricondotto in prima istanza a quello, che pure viene legittimamente evocato, dei costi della politica.

sul cosiddetto pareggio di bilancio, che anche noi abbiamo proposto. Ebbene, quelle decisioni ci hanno fatto comprendere una cosa: come l'architettura istituzionale di un Paese abbia a che fare, molto da presso, con la sua salute economica.

a salvaguardare la salute economica degli Stati. Nessuno nega, dunque, che esista un problema di aggiornamento delle nostre istituzioni e che tale aggiornamento abbia a che fare anche con i costi della politica. Questo è il modo giusto di porre la questione. Cari colleghi, noi abbiamo una buona Costituzione, frutto di un alto compromesso che si fece nel dopoguerra, ma è l'ultima Costituzione di prima generazione che ancora resiste in Europa. Si riferisce ad un tempo nel quale il mondo andava in maniera diversa, i meccanismi della globalizzazione erano differenti e i tempi della decisione erano diversi. Non c'è dubbio

perché se si cambia il sistema della legge elettorale passando, ad esempio, come voi dell'IdV chiedete, a un sistema di collegi, è necessario tutto il territorio nazionale venga coperto da collegi che possano reggere il meccanismo uninominale al quale con la vostra iniziativa referendaria fate riferimento.

tende a passare da un sistema di liste ad un sistema di collegi uninominali. Allora, vogliamo tener conto di tutto ciò è vogliamo provare a a legare la riduzione del numero dei parlamentari a una ridefinizione della rappresentanza e delle funzioni dei due rami del Parlamento? Credo che se vogliamo veramente cercare di incidere in maniera non demagogica ma seria sui costi della politica questo tentativo debba essere esperito. Non possiamo

a ridurre il numero dei parlamentari senza agire sulle funzioni delle due Camere e senza considerare le conseguenze del *referendum* in realtà

Queste, colleghi, non sono scuse per mantenere la situazione attuale. Siamo assolutamente consapevoli che non abbiamo né la possibilità né il tempo - non ce l'ha il Paese - di buttare la palla in calcio d'angolo o in fallo laterale. Siamo assolutamente consapevoli che su questo ci giochiamo una partita fondamentale Vorremmo solamente non ridurre le istituzioni a un osso da lanciare a qualcuno che ci pone il tema dell'antipolitica e ridurre tematiche fondamentali che hanno appassionato generazioni e generazioni, iniziando dai Padri costituenti, problemi che ineriscono solamente una questione di costi. I parlamentari vanno ridotti, ma perché vanno ammodernate le nostre istituzioni. le nostre istituzioni. La riduzione del numero dei parlamentari non è solamente una questione di costi, e qualcuno in passato l'ha sperimentato, arrivando persino all'abrogazione dell'istituto parlamentare. Non è questa la strada. La strada è legare questo tema ad un grande progetto di cambiamento. Colleghi, un grande liberale del dopoguerra, Vittorio De Caprariis, diceva che le istituzioni sono anche passioni. Poi è arrivato il tempo degli ingegneri costituzionali - a cui qualcuno di voi ha fatto riferimento - e parte di quella passione si è persa. Vorremmo evitare di inaugurare un'altra stagione nella quale il costo di un parlamentare viene equiparato al problema del costo di una bistecca o del riso in bianco nel ristorante del nostro Senato.

Signor Presidente, intervengo solo per esprimere con chiarezza il mio pensiero sulla richiesta avanzata dal presidente Belisario. Per un profilo tecnico, debbo ricordare che il disegno di legge n. 2891 è stato presentato il 5 settembre 2011 e annunciato nella seduta pomeridiana del 6 settembre. Il 7 settembre è stato assegnato in sede referente alla Commissione affari costituzionali che, nello stesso giorno, ne ha iniziato l'esame. I relatori, senatori Boscetto e Bianco, lo hanno infatti illustrato insieme agli altri disegni di legge di analogo contenuto.

dopo la pausa estiva, che poi non c'è neanche stata, e quindi lo abbiamo anche anticipato. Detto questo, mi rendo conto che, dietro la richiesta della dichiarazione d'urgenza, non vi è solo un fatto tecnico ma viene posta anche una questione quella di cui mi pare si sia dibattuto per tutta la mattinata in quest'Aula. Voglio dire che il metodo di lavoro che pare possa andare avanti è convincente, se si realizza una sola condizione: che, alla luce del disegno di legge che il Governo presenterà e di quelli già presentati dai Gruppi politico-parlamentari su riforme della Costituzione, si possano trovare questioni che si approvano con una maggioranza superiore a quella dei due terzi, se vogliamo che qualcosa entri in vigore già dalla prossima legislatura. Tutto il resto, infatti, sarebbe una finzione poiché, dovendo celebrare un *referendum* che inevitabilmente dovrebbe essere fissato dopo dopo le elezioni, se si va a scadenza naturale, nulla entrerebbe in vigore prima del 2018. Dobbiamo dire questo con grande franchezza perché gli italiani

la dichiarazione di urgenza, per quanto mi riguarda mi asterrò dal partecipare alla votazione. Non ritengo infatti di poter andare più veloce di quanto già fatto e quindi non posso votare la dichiarazione d'urgenza. Non vorrei però che, votando contro da presidente della Commissione affari costituzionali, qualcuno potesse pensare che dietro il voto contrario si nascondano altri progetti che francamente non ho, anche perché non ho la disponibilità dei lavori della Commissione, che sono nelle mani dei Gruppi parlamentari che si esprimono nell'Ufficio di Presidenza all'unanimità o nella Commissione plenaria a maggioranza. Per queste ragioni, non parteciperò

senatrice Poretti. So di non dare un dispiacere al senatore Li Gotti nel confermargli che non sono nel pieno possesso delle mie capacità intellettive, perché se lo fossi avrei capito il motivo per cui l'Italia dei Valori, unico vero partito di opposizione, chiede una procedura di urgenza non per il conflitto di interessi, ma per un qualcosa che si tratta la settimana prossima, e del perché - se il problema dovesse essere quello della lotta alla casta - non ha chiesto l'urgenza per l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti,

occupati per tre ore. Anzi, spero che qualcuno, esperto nei processi cognitivi, studi nel dettaglio queste tre ore di dibattito, perché veramente se ne può trarre una conclusione degna delle migliori pubblicazioni scientifiche! *(Applausi dai Gruppi

che sicuramente entreranno in un Parlamento nominato dalle oligarchie partitocratiche e sono attaccati ai poteri forti! *(Applausi dai Gruppi PdL, che voi non avete voluto, con la vostra emergenza, mettere all'ordine del giorno del nostro dibattito, e di oggi, e di tutti gli anni in cui siete rimasti a fare l'opposizione a questo regime - che comunque non chiamate così - e che sono quelli rappresentati dal cattivone Silvio Berlusconi, che comunque continua a mantenere tutti i suoi conflitti di interessi perché nessuno si mette in animo di porre all'ordine del giorno il problema da affrontare, e che va affrontato, che è quello Allora, pur condividendo totalmente il merito della dichiarazione del presidente Bianco, votiamo contro questa proposta. - capisco che chi è tutte le sere in televisione come l'onorevole Di Pietro deve avere qualcosa di più da dire, altrimenti viene a noia anche a chi lo intervista e a se stesso - sicuramente diciamo no ad un voto che certifichi la professionalizzazione dell'anticasta, perché questo è: si fanno tanti bei soldi certamente anche esercitando questo tipo di opposizione. Ma non con il voto della senatrice Poretti e del senatore Perduca!

come sappiamo la speciale procedura che stiamo espletando, prevista dall'articolo 77 del nostro Regolamento, prevede l'attribuzione del carattere di urgenza ad uno specifico disegno di legge. il presidente Belisario ha chiesto il pronunciamento sul disegno di legge presentato da lui stesso e dal suo Gruppo. il 16 settembre 2011 è stato presentato

e, anzi, di contenuto sostanzialmente analogo, se l'oggetto della votazione attrae o meno tutti i disegni di legge presentati su questa materia, come io ritengo debba essere. Senatore Legnini, la richiesta, fatta dal senatore Belisario, della dichiarazione

Questa è una richiesta specifica.

sembra arrivare per ultimo perché, quando abbiamo capito che forse vi era la volontà di portare a compimento almeno la riduzione del numero dei parlamentari, lo abbiamo stralciato di riforma più organica che avevamo presentato anche noi qualche anno fa.

della collega Finocchiaro. Pertanto, io ritengo che, vista anche la dichiarazione di intenti del proponente stesso, che si debba rispettare quanto la Commissione ha già fatto.

Presidente, alla luce delle dichiarazioni che si sono svolte da ultimo e considerando che da questa mattina parliamo esattamente di questa materia, noi senatori del Terzo Polo dichiariamo che non parteciperemo ad una votazione che ci pare incomprensibile e totalmente priva di senso, alla luce delle decisioni che sono state assunte in

Abbiamo convenuto che entro quaranta giorni - il senatore Quagliariello ha raccolto la proposta che noi abbiamo fatto - ci si ritrovi in Assemblea a valutare esattamente il progresso delle norme di modifica costituzionale che sono all'esame del nostro e dell'altro ramo del Parlamento. Abbiamo tutti convenuto sul fatto che è impossibile procedere con la riduzione del numero dei parlamentari se non contemporaneamente, alla modifica alla modifica della legge elettorale e se non in un contesto che chiarisca le funzioni del Senato, perché non sarà più il Senato paritario con la Camera dei deputati. È chiaro allora che questa questa maniera di chiedere delle misure spot per mettersi le penne del pavone non ha alcun senso politico. Noi pertanto non partecipiamo alla votazione. Presidente, anche alla luce degli interventi dei colleghi, le chiedo espressamente di voler adottare una interpretazione che sia la più logica e coerente della norma regolamentare contenuta nell'articolo 77, nel senso che non si può evidentemente dichiarare la procedura d'urgenza su un disegno di legge contenente le modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, presentato un mese fa, quando ce ne sono altri presentati tre anni fa, tra cui il nostro, e soprattutto allorquando la Commissione affari costituzionali ha già predisposto un testo unificato, nel quale penso sia confluito anche il testo

conseguentemente alla richiesta del presidente Belisario, il pronunciamento d'urgenza sui disegni di legge, vertenti in materia di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Non credo che possa essere disposto diversamente. La sollecito, pertanto, ad adottare una decisione in tal senso. In effetti mi comunicano gli Uffici che ci sono dei precedenti per cui l'abbreviazione dei termini, sulla base della richiesta del proponente, si estende ai disegni di legge unificati. In questo senso il presidente Belisario, che pure aveva fatto una richiesta specifica

ha richiesto l'abbreviazione dei termini su tutti i disegni di legge unificati. Per questo motivo è chiaro che la decisione riguarda il testo unificato in discussione in Commissione.

fatte sulla virtualità di questa discussione alla luce dell'ottimo lavoro che la 1a Commissione sta facendo: sta infatti lavorando, ha posto dei termini e vi è un calendario preciso. Quindi, la richiesta d'urgenza ha scopi puramente propagandistici e inutili. Alla luce del fatto che lei ha annunciato che comunque la richiesta logicamente riguarda l'insieme dei disegni di legge, il nostro Gruppo si asterrà nella votazione, perché non vuole partecipare ad una commedia degli inganni in cui qualcuno potrebbe dire che taluni sono favorevoli ad una certa scelta e altri sono contrari. Non condividiamo questa procedura che inutilmente si sovrappone all'ottimo lavoro che la Commissione sta facendo. Quindi, ci asterremo.

sul disegno di legge Belisario o di tutti disegni di legge di fatto all'attenzione in questo momento della 1a Commissione vuol dire allungare i tempi. Siamo già in fase di presentazione degli emendamenti. Dalla settimana prossima si votano gli emendamenti in Commissione. La dichiarazione d'urgenza non vuol dire bypassare la Commissione; comunque bisogna riaprire una discussione generale e bisogna fissare nuovamente i termini per la presentazione degli emendamenti.

Dopo l'intervento del presidente Gasparri ho chiesto al presidente Belisario e anche al senatore Rutelli se intendevano procedere con la votazione di questa richiesta, perché è evidente che una via poteva essere quella,

Presidente, sentendola parlare mi era venuto

l'istituto dell'astensione, in quanto con tale istituto ci si sottrae alla responsabilità e si cerca una mediazione; ma la mediazione si può cercare solo e soltanto sulle soluzioni, non già sui principi.

sia per il lavoro che stanno svolgendo i consiglieri regionali della lista Bonino-Pannella in Regione Lazio, sia per l'ottimo lavoro che sta portando avanti il compagno radicale Massimiliano Iervolino, che ha scritto un libro sull'argomento dal

appunto un ottimo lavoro. La Relazione conclusiva ha evidenziato in modo puntuale le criticità che, negli ultimi undici anni, non hanno trovato soluzione. Il testo licenziato dall'organismo parlamentare ha ben indicato le responsabilità, al riguardo davvero *bipartisan*: infatti, né il centrosinistra, né il centrodestra hanno saputo e voluto programmare un ciclo dei rifiuti conforme Il Lazio non è la Campania semplicemente perché nella Regione della Capitale esiste la discarica più grande d'Europa, una discarica illegale che va contro tutte le leggi nazionali ed europee. Il commissariamento non ha risolto nulla. Questo strumento emergenziale non ha raggiunto lo scopo principale, quello di redigere un piano rifiuti conforme alle direttive dell'Unione europea, ma è servito solamente ad autorizzare volumetrie straordinarie di discariche: questo è il nostro parere e, da quello che leggiamo, anche quello della Commissione bicamerale. Il 30 giugno 2008 finiva la gestione straordinaria sui rifiuti: continuava dal 1999, doveva durare un solo anno e in quei dodici mesi si doveva stilare un piano. Invece ci sono voluti nove anni per uscire dal commissariamento, e ancora oggi il piano non c'è. Per legge, entro il 2003 la raccolta differenziata doveva raggiungere il 35 per cento, e per centrare questo obiettivo furono stanziati 64 milioni di euro. Gli ultimi dati ufficiali, che risalgono al 2008, dicono che non si supera il 20 per cento. Nella regione Lazio la produzione di rifiuti solidi urbani (dati rapporto rifiuti ISPRA 2008) è stata nel 2007 di 3.359.554 tonnellate, con una produzione *pro capite* di 604 chili per abitante per anno, con un aumento di circa il 14 per cento rispetto al 2003. Di questa quantità enorme di rifiuti, circa l'83 per

la nomina del prefetto Pecoraro come commissario. Questo dovrà prendere quelle decisioni che né il sindaco di Roma, né la presidente del Lazio, il cui comportamento è da definirsi molto grave, anche perché i poteri speciali nel nostro Paese hanno sempre creato solo altri disastri, Negli ultimi dieci anni la percentuale di raccolta differenziata nella regione Lazio è rimasta abbastanza costante senza subire notevoli variazioni, a dimostrazione che la cultura della discarica è stata predominante per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dai dati sopra riportati si evince che la stragrande maggioranza dei rifiuti solidi urbani viene conferita in uno dei dieci invasi presenti nel territorio. È bene ricordare che la direttiva 1999/31/CE dell'Unione europea stabilisce che in discarica possono entrare solo rifiuti pretrattati, cioè quelli depurati dalla raccolta differenziata.

per via di proroghe annuali generalmente contenute nelle leggi finanziarie. Roma non è Napoli grazie a queste proroghe annuali, ma se il Parlamento rispettasse le direttive europee in materia e, quindi, le leggi che l'Italia si è data, nella Capitale ci sarebbero tonnellate e tonnellate di rifiuti per strada. Quindi L'illegalità dei conferimenti è sotto gli occhi di tutti e questa produce disastri ambientali. Infatti, è notizia degli ultimi giorni che la procura di Roma ha aperto un'inchiesta relativa a quattro morti sospette di cittadini che vivevano vicino la discarica di Malagrotta. L'ultimo piano dei rifiuti della Regione Lazio risale al 2002. In materia di rifiuti è molto importante la programmazione, ma la classe politica della Regione Lazio non ha saputo ottemperare ai suoi compiti. si può dichiarare, senza timore di essere smentiti, che i Governi che si sono succeduti, al di là dei colori politici, sono complici di questa allarmante situazione. Il commissariamento durato tanti anni non è servito a uscire dall'emergenza,

grado di precisione sufficiente per assicurare la piena efficacia della direttiva 1975/442/CE» e non consente di «individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi». Di conseguenza, non avendo l'Italia ottemperato alla sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha deciso di procedere con una seconda lettera di messa in mora. A tale messa in mora la nuova Giunta regionale in carica, guidata dalla presidente Polverini, ha risposto approvando un piano che, è bene sottolinearlo, non ha ancora ricevuto il consenso del Consiglio regionale ma, per ora, solo l'accettazione

Il piano regionale dei rifiuti della giunta di centrodestra non risolve i problemi che anche la Commissione bicamerale ha evidenziato. Come detto in apertura, Roma non è apparentemente nella stessa situazione di Napoli grazie alla discarica di Malagrotta, ma i problemi delle due grandi città sono simili: bassa percentuale di raccolta differenziata, *deficit* di impianti di trattamento meccanico-biologico e di impianti di compostaggio, mancanza di mercato delle

Per troppo tempo, in modo assolutamente *bipartisan*, la politica della Regione Lazio non ha voluto avviare un ciclo virtuoso dei rifiuti e ha continuato a conferire più dell'80 per cento dei rifiuti solidi urbani nelle discariche. In queste - è bene chiarirlo, come ha già fatto la Commissione bicamerale - si conferisce anche CDR di bassa qualità e parte della raccolta differenziata, altrettanto di bassa qualità qualità o non trattata in impianti adeguati. La discarica di Malagrotta è un problema soprattutto ambientale: si stima che negli anni siano stati sotterrati circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti e, come conseguenza, c'è un inquinamento elevatissimo nella zona. A confermare questa allarmante situazione è l'ultimo rapporto dell'ISPRA, che solo ieri abbiamo potuto leggere; questo lavoro scientifico ha dimostrato, per l'ennesima volta, il disastro ambientale che i cittadini di Ponte Galeria e di Massimina devono subire. I controlli sono stati, e continuano ad essere, fallaci. La popolazione che vive a ridosso della discarica ha più volte denunciato l'inoperosità delle giunte, di centro, di destra e di sinistra, nel risolvere questo grave problema. L'Europa ha aperto una procedura di infrazione contro la discarica, proprio per i motivi che ho denunciato in apertura, cioè l'assoluta illegalità del conferimento di rifiuti non trattati. Malagrotta va chiusa perché è un mostro che uccide l'ambiente. Nella Relazione della Commissione bicamerale c'è la strada giusta da seguire (che però finora non è stata portata avanti dai governi regionali): riduzione e riciclo dei rifiuti e recupero di materia e di energia, in perentorio ordine di priorità. Invece il Lazio ha un sistema basato principalmente sulle discariche e sugli inceneritori, senza avere una riduzione degna di questo nome e una raccolta differenziata da Paese civile. Questi sono anche gli obiettivi che i tanti comitati di cittadini chiedono alla propria amministrazione, che - è bene dichiararlo di nuovo - purtroppo non si è voluta assumere le proprie responsabilità e ha delegato al prefetto decisioni importanti che dovevano essere prese da chi è stato eletto per questo, cioè la presidente Polverini e il sindaco Alemanno.

Presidente, la risoluzione n. 1 e la Relazione da cui è ricavata, che è stata approvata dalla Commissione bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, fotografano la situazione di una Regione *borderline*. Dal punto di vista della gestione dei rifiuti, il Lazio è sull'orlo di un precipizio: anzi, penso sia sull'orlo di due precipizi. Il primo dipende

il primo precipizio di fronte al quale i cittadini del Lazio si trovano è rappresentato dall'incapacità di smaltire i rifiuti che si producono quotidianamente. La discarica di Malagrotta sta per essere chiusa; è in corso un balletto, anche abbastanza irresponsabile, tra la Regione e il Comune di Roma, per quanto riguarda la localizzazione di un nuovo sito: il Comune rifiuta di localizzarlo nel proprio territorio (ricordo che Roma è il più è il più grande Comune agricolo d'Italia e ha un territorio molto vasto) e la Regione insiste per questa scelta. Comunque, ad oggi non c'è un'alternativa chiara e definita

che ha dato luogo a moltissime inchieste della magistratura, a moltissime polemiche e denunce da parte delle associazioni ambientaliste. Questo è il primo precipizio davanti al quale ci

delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti che, come è noto, in Italia sono molto rilevanti. Anche da questo punto di vista, il Lazio è una Regione *borderline*, dove già da tempo è entrata con prepotenza la criminalità organizzata: forse è l'unica Regione italiana dove lavorano, non a braccetto, naturalmente, ma contemporaneamente tutte e tre le grandi organizzazioni criminali d'Italia: la camorra, la mafia e la 'ndrangheta. In particolare, nella parte meridionale del Lazio, questa situazione ha raggiunto livelli drammatici. Cito per tutti il caso della discarica di Latina, quella di Borgo Montello, che incombe su quel territorio anche fisicamente su un grande campo rom, e che si sta cercando faticosamente di risanare, finora senza risultati totalmente soddisfacenti. Su tale discarica incombe anche fisicamente la presenza del clan dei casalesi, proprietari di terreni a poche centinaia di metri dal sito della discarica. La discarica di Borgo Montello è già stata al centro anch'essa di inchieste della magistratura per possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Questa è oggi la situazione del Lazio. È utile il lavoro fatto dalla Commissione è utile la risoluzione, ma lo è soltanto se tutti quelli che hanno responsabilità di decisione capiscono che manca poco tempo per evitare che il Lazio cada definitivamente sia nel precipizio di tipo napoletano dell'impossibilità di mettere da qualche parte i rifiuti solidi urbani che si producono ogni giorno, sia nell'altro precipizio, ossia in quello delle ecomafie e del loro strapotere. Per il momento le cose scritte nel documento in esame sono certamente un atto di responsabilità, ma il vero atto di responsabilità saranno chiamati chiamati a compierlo nelle prossime settimane - nemmeno, credo, nei prossimi mesi - la Regione Lazio e il Comune di Roma, che hanno chiesto, io credo giustamente, che finisse la gestione commissariale, e che adesso devono dimostrare di essere in grado di fare quello che si fa in tutta Europa e in gran parte d'Italia: raccolta della differenziata almeno al 50

Da anni le associazioni ambientaliste, ma non solo, chiedono inutilmente che finalmente nel codice penale italiano vengano inserite le fattispecie di reati connessi in particolare

che un gesto apparentemente semplice, ma che si aspetta da 15 anni, sarebbe un primo modo concreto per dimostrare che quelle scritte dentro la risoluzione condivisa non sono soltanto parole.

facoltà. COSENTINO *(PD)*. Signor Presidente, ho qui la fotocopia di un fonogramma che il direttore del Servizio dell'Assemblea ha inviato all'onorevole Elio Vito sollecitando la risposta a un'interrogazione: banalità, direi. Tuttavia è curioso verificare che la data del sollecito è il 29 settembre 2010. Domani sarà passato un anno da un sollecito con il quale il Senato chiede risposta ad un'interrogazione. Io non chiedo di sollecitare nuovamente perché non ho nessuna fiducia in un Governo che si dimostra così maleducato. Chiedo invece al Presidente dell'Assemblea di sapere quante sono le interrogazioni presentate nel corso della legislatura che non hanno ricevuto risposta dal Governo. Mi pongo infatti la domanda del perché la Presidenza del Senato non sia in grado di garantire il rispetto delle prerogative del Parlamento. senz'altro preparato un quadro della situazione.

se sia stata soddisfatta o meno. Il quadro delle interrogazioni che sono state presentate e quanto è stato disposto può essere fatto, e sarà fatto, e questo, quindi, senatore Cosentino, l'avrà. Per il resto, penso che ci siano problemi che non sono semplicemente legati alla volontà del Senato o dello stesso Governo. Il problema è che noi abbiamo dei meccanismi regolamentari, a differenza di altri Parlamenti

Signor Presidente, questa mattina a Genova sono di nuovo scesi in piazza gli operai di Fincantieri. Lo avevano già fatto a maggio, con l'appoggio di tutta la cittadinanza. si erano riuniti anche con gli operai di cantieri di altre realtà italiane. C'era stata una presa di posizione del Governo che aveva richiesto all'amministratore delegato di ritirare il piano industriale che era

è stato firmato un accordo di programma per il «ribaltamento a mare» e, il Governo si è assunto l'impegno di versare 70 milioni; in realtà, per ora, pare che ne siano disponibili solo 50 che non sono ancora stati destinati,

a rispondere in qualche modo. Io conosco bene il settore militare: so che la Marina, senza le dieci FREMM previste non è in grado di svolgere il proprio ruolo. Quattro sono già state ordinate, ma delle altre non si ha traccia.

consistente. Parlo delle commesse militari perché è la prima cosa che il Governo potrebbe fare, ma potrebbero essercene altre. Ad esempio, si potrebbero prevedere incentivi per rinnovare la flotta mercantile. Ciò che chiedo è che nel «decreto sviluppo» si tenga conto di queste cose, altrimenti quando parliamo di sviluppo nel nostro Paese di cosa stiano parlando se non diamo lavoro e non diamo prospettive ai cantieri navali, che sono un fiore all'occhiello della manifattura italiana? Chiedo dunque, per favore, alla Presidenza del Senato

mi faccio personalmente carico di rappresentare al Governo, nelle persone del Ministro della difesa e del ministro Romani, le necessità e le richieste che vengono dalla città Fincantieri è un'importante realtà e come tale va difesa; è una realtà anche qualitativa, non solo quantitativa, fiore all'occhiello dell'industria italiana, e credo che sia davvero doveroso fare in modo che non ci

all'azienda e alle sue maestranze.

quella cricca di soggetti privati come Moody's, Standard & Poor's e Fitch che continuano ad emettere pagelle ad orologeria nonostante non siano state richieste, condizionando ogni giorno i corsi dei cosiddetti mercati, dai quali dipendono le sorti di Governi e Stati sovrani, che almeno si sono conquistati, nei sistemi democratici, la legittimità popolare. Martedì scorso, mentre tutti aspettavano le pagelle da parte di Moody's, è arrivata quella di Standard & Poor's che ha declassato l'Italia da A+ ad A. Faccio notare al Parlamento che alla data di oggi Standard & Poor's, come le altre consorelle Fitch e Moody's, non risultano iscritte, ai sensi dei regolamenti europei, all'ESMA, una delle tre autorità di vigilanza, con sede a Parigi, rue de Grenelle, 103. Nonostante avessero fatto richiesta, non hanno superato l'esame,

alla data di oggi né Moody's, né Fitch, né Standard & Poor's, risultavano iscritte. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione dicendo anche se non conosciamo le motivazioni di questa bocciatura, riteniamo siano state escluse per conflitti di interesse nel loro azionariato. Standard & Poor's *-* ad esempio - è partecipata di un fondo che gestisce un patrimonio di 3.000 miliardi di dollari, ripeto 3.000 miliardi di dollari, BlackRock (tradotto: roccia nera),

ha messo in cantiere i funerali dell'euro e dell'Europa. Io mi rifiuto di partecipare e quindi, come sempre,

fatta di fondi speculativi, banche e banchieri centrali i cui comportamenti - mi consenta - sono ancora peggiori dei criminali seriali che operano nell'ombra e nell'illegalità, emettendo montagne di derivati, OTC, SWAP, denaro dal nulla, pari a 700.000 miliardi di dollari contro un PIL del mondo, che misura la fatica degli uomini, di 55.000 miliardi di dollari. Bisogna porre fine a questa speculazione a danno della povera gente, dei popoli, dei risparmiatori e degli stessi Stati. Ieri ne abbiamo parlato in Commissione finanze. Adesso vedremo vedremo se presentare una risoluzione o una mozione. L'Europa per fortuna ha battuto un colpo con la Tobin *tax*, ma bisogna ribellarsi. È la politica che detta le regole e gli oligarchi eseguono, e non il contrario! Siamo sotto ricatto dei mercati,

Dalle nostre parti, caro Presidente, si dice che «a settembre l'uva è matura e il fico pende». Siamo pronti a raccogliere i frutti di un'estate che si spera sia andata bene.

proposta dai poteri forti testé ricordati dal senatore Lannutti e dichiarata esclusivamente di fronte alla stampa, ma non di fronte alle Commissioni competenti, dal Ministro dell'interno. nel settembre 2009 abbiamo svolto un dibattito in Commissione affari costituzionali, e di questo si parlò. Furono distribuiti dei dati in cui si certificava come negli ultimi tre anni fossero diminuiti gli incidenti dentro e fuori dagli stadi.

stamane abbiamo avuto tre ore di dibattito sul nulla, nel pomeriggio si discuterà dell'Alzheimer, credo che ci siamo, anche dal punto di vista del merito della questione. Occorrerebbe però sapere perché non si vuole dare una risposta - che a me è stata data personalmente al bar, e quindi non ha potuto essere inclusa negli atti su che cosa sia questa benedetta tessera del tifoso, anche perché ci viene detto quotidianamente che è obbligatoria, e noi stiamo limitando i diritti costituzionali degli italiani relativamente relativamente a qualcosa che certo non necessariamente interessa tutti, ma che è la libertà di movimento. Infatti, si preclude la possibilità di mettersi a sedere in un settore dello stadio se non si ha questo fantomatico tesserino, i cui dati includono addirittura ciò che è al centro del *file* individuale del casellario giudiziario. Anche questo è un altro esempio di come la legge, da una parte, addirittura non esista, ma dove esiste (e qui (e qui parlo delle regole relativamente alla *privacy* individuale) venga calpestata. Dopo due anni di pazienza, io credo che sia il caso di risollecitare questa interrogazione parlamentare per avere una parola. Mi accontento anche di un Sottosegretario, non c'è bisogno